L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Signor Presidente, è una mattinata difficile per tutti noi. L'attacco della Russia all'Ucraina è di una gravità inaudita. Riteniamo necessario che il Senato voti la condanna ferma e unanime dell'attacco russo e dell'invasione militare. Non ci possono essere spazi per distinguo o per ambiguità. Per questo chiediamo che il presidente Draghi, dopo le riunioni di oggi nei diversi ambiti della NATO e dell'Unione europea,

voglio riprendere le parole del Papa di qualche giorno fa, quando ha detto che l'umanità, che si vanta di andare avanti nella scienza e nel pensiero, va indietro invece nel tessere la pace e questo ci fa vergognare tutti.

dalla voce del presidente Draghi quali siano le scelte, le reazioni e le misure che l'Italia intende adottare insieme ai *partner* europei e internazionali, nella speranza che, almeno questa volta, l'Unione europea e l'Occidente sappiano far sentire forte la loro voce.

dell'Ucraina. Diamo massimo sostegno al presidente Draghi affinché venga data una risposta comune da parte degli alleati. Serve un Occidente forte, compatto e unito. naturalmente è che cessino subito le ostilità e si torni sulla linea della diplomazia e del dialogo, che è la via principale per risolvere i conflitti. Cito, a tal proposito, una dichiarazione fatta dall'ex segretario di Stato americano Richard Nixon il 5 marzo del 2014, l'Ucraina deve rappresentare un ponte tra l'Occidente e la Russia e non un avamposto dell'una contro l'altra e viceversa.

mettere in evidenza che la diplomazia italiana, che ha sempre avuto un ruolo importante e una lunga tradizione nei

Presidente-UDC condanna la guerra ed è per la pace. Questo è il momento di essere tutti uniti per un solo obiettivo: la pace, la pace. Tutto il mondo occidentale deve compattarsi per far sentire forte la propria voce in maniera univoca, la voce di una comunità internazionale che deve lavorare per questo. Quindi, chiediamo anche noi che il presidente Draghi venga in quest'Aula a condividere le idee del Governo con il Senato, che darà ogni contributo possibile per il raggiungimento del valore

ma anche - palesemente - del diritto internazionale. Ecco perché siamo al fianco del nostro Governo. L'operato tenuto in queste settimane è quello giusto: al fianco dell'Alleanza atlantica e dell'Europa, con una voce dell'Occidente chiara nel tentativo di evitare il conflitto, ma anche nell'intenzione di assumere una decisione ferma e risoluta contro quest'*escalation* di violenza. violenza. Ci uniamo pertanto anche noi alla richiesta che il presidente del Consiglio Draghi venga a riferire in Aula dopo che l'Unione europea abbia assunto delle risolute decisioni in merito alle sanzioni da adottare,

L'Italia è a fianco della democrazia, dei diritti e dei valori democratici insieme all'Europa e alle forze atlantiche.

perché si torni indietro e si interrompa un'*escalation* che rischia di essere veramente drammatica per tutta l'Europa. Siamo vicini in questo momento alla popolazione civile che, ancora una volta, rischia di dover pagare in prima persona con morti e feriti. *(Applausi)*. UV))*. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo Per le Autonomie condanna fermamente l'atteggiamento aggressivo e criminale di Putin e della Russia verso l'Ucraina. Se ci fosse bisogno di precisarlo, si trattava non solo di un atteggiamento autonomista di Putin verso alcuni territori dell'Ucraina, ma anche di un progetto ben più ampio e più aggressivo, che rischia di portare la guerra in Europa dopo settant'anni. Naturalmente, nel sottolineare tutta la nostra solidarietà al popolo ucraino e al suo Governo, anche noi concordiamo pienamente con la richiesta di audire al più presto il presidente Draghi.

registrato. La Presidenza si unisce ai sentimenti di condanna espressi unanimemente dal Senato della Repubblica e all'auspicio di pace con giustizia che viene da parte di tutti i i Gruppi. Riferirò immediatamente la richiesta avanzata da numerosi Gruppi, o da tutti, di audire al più presto, quando si riterrà più opportuno, il presidente Draghi.

ci troveremo tra qualche minuto al quarantesimo voto di fiducia di questa maggioranza veramente ipertrofica; se non veramente ipertrofica; se non fosse che Fratelli d'Italia è l'unico partito a sostenere la discussione generale

dalla sanità ad altri, che attengono a passaggi importanti della vita quotidiana della nostra Nazione; se non fosse che

da quando siedo su questo scranno e che, nel discorso di insediamento del Presidente della Repubblica, è stata additata

nelle Commissioni competenti, perché ce ne sarebbe stato il tempo e sicuramente ci sarebbe stata anche la volontà, da parte nostra, come partito di opposizione,

invece appello, in questo mio intervento, al senso di rispetto delle istituzioni che so essere presente in tanti colleghi, in ognuno di voi, affinché veramente tutto ciò non si

Oggi siamo in presenza di numerose emergenze, fra le quali paradossalmente quella sanitaria sembra essere la meno preoccupante. Abbiamo alle porte un'emergenza geopolitica che fino adesso i nostri Capigruppo hanno trattato. Abbiamo alle porte una crisi economica drammatica. Credo e spero che il Parlamento, in un sussulto di dignità

solitamente intervengo in Aula solo su provvedimenti che riguardano la Commissione a cui appartengo, e quindi per parlare di ambiente. Da quando, però, c'è questo Governo intervengo poco, perché l'ambiente è stato di fatto abrogato. Oggi, invece, intervengo per ribadire nuovamente che il Parlamento è stato totalmente messo al tappeto da Draghi e vorrei invitarvi a fare un minuto di riflessione, prima che sia troppo tardi. Tanti si sono spesi in quest'Aula l'altro giorno per difendere le prerogative parlamentari reclamate dall'ex Presidente del Consiglio Renzi e non vi accorgete che ci stanno togliendo sostanzialmente la funzione principale del parlamentare, sancita dalla nostra Costituzione. Questo Governo sta smantellando ogni prassi, ogni regola democratica e anche ogni parvenza di esse. Più volte si è discusso dell'arroganza dei Governi, spessissimo di quello attuale a cui orgogliosamente non ho dato la mia fiducia, che ha esautorato il ruolo del Parlamento con l'abuso spropositato dei decreti-legge. Più volte abbiamo lamentato il loro utilizzo e soprattutto l'uso della fiducia sui decreti, che ha raggiunto la sua massima perversione con la sistematica apposizione della doppia fiducia in entrambe le Camere sul medesimo provvedimento. Così era rimasta soltanto l'apparenza del Parlamento, dando la possibilità alle Commissioni competenti almeno dell'espressione di un parere. Si trattava solo di apparenza, però, perché capite bene che un lavoro vero e serio su leggi che vanno a cambiare la vita delle persone non può essere svolto in due o tre giorni, ma richiede tempo: il tempo necessario per un confronto, per ascoltare, per approfondire. Oggi possiamo dire che non è rimasta nemmeno l'apparenza di quello che era il Parlamento: siamo arrivati al culmine di un'indecenza divenuta, appunto, prassi consolidata. In qualità di Presidente della Commissione ambiente, ieri mi è stata comunicata l'assegnazione - per l'espressione del parere - del decreto-legge cosiddetto milleproroghe, il cui esame alla Camera si è concluso il 22 febbraio, con la questione di fiducia ovviamente.

minuti per essere pronti per le 9,30 di stamattina. *(Applausi)*. Avete convintamente votato per eleggere nuovamente il presidente Mattarella per poi non dare minimamente ascolto alle sue parole? Pochi giorni fa lo stesso Presidente della Repubblica nel suo discorso ha «Un'autentica democrazia prevede il doveroso rispetto delle regole di formazione delle decisioni, discussione, partecipazione». Spero vi rendiate conto che qui si tratta non di maggioranza o di opposizione e nemmeno della necessità o meno di un provvedimento, ma della stessa esistenza e utilità della funzione delle Camere e dei loro componenti. Continuando in questo modo state abdicando alla vostra funzione; vi state dichiarando inutili, forza. Lo ripeto per essere chiari affinché rimanga agli atti: il Parlamento non esercita più la sua funzione legislativa e neanche quella sacrosanta di controllore del Governo. Ai parlamentari, a tutti noi viene negato il diritto di esercitare le nostre funzioni, quelle per cui siamo stati eletti. Ora o pretendiamo insieme - maggioranza e opposizione - il rispetto del Parlamento oppure saremo costretti, quando incontreremo un cittadino o un'impresa, a rispondere che noi come parlamentari non abbiamo il diritto neanche di fiatare, perché siamo in una vera e propria dittatura. Spero che possiate davvero riflettere su quello che sta succedendo: è un qualcosa che non fa bene a noi come rappresentanti dei cittadini, ma di certo non fa bene al Paese. Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, se non ci fossero apprezzabili circostanze nel grave quadro internazionale che si è determinato, anche oggi sarebbe andata in scena la triste prassi del fuggi fuggi del giovedì. Siamo al cospetto di un provvedimento *omnibus* per sua natura, il milleproroghe, che si avvia mestamente verso un nuovo voto di fiducia. Lo ha detto il collega Zaffini: saremo al cospetto del quarantesimo voto di fiducia in un anno del Governo Draghi, che si avvia a battere tutti i *record*, stracciando perfino quelli che avremmo ritenuto insuperabili del Governo Monti. La maggioranza rinuncia a circa quattr'ore di discussione generale. Tutti hanno applaudito il discorso del presidente Mattarella quando ha richiamato al rispetto delle prerogative del Parlamento tra coloro che applaudivano, ci sono gli stessi parlamentari che oggi rinunciano alla discussione generale che nelle scorse settimane hanno applaudito parimenti ai rappresentanti dei Gruppi che invitavano a consegnare l'intervento in dichiarazione di voto. Se non siamo innanzitutto noi a essere coerenti con il ruolo che il popolo ci ha affidato, eleggendoci quali loro rappresentanti, da chi vogliamo che venga fatta rispettare la nostra alta funzione di rappresentanza della Nazione? Bisogna invocare il rispetto per il Parlamento, certamente, ma il rispetto nessuno ce lo può dare se non siamo capaci innanzitutto noi. Si continua con il metodo della decretazione d'urgenza, in molti casi creativa. Stiamo ad assistere, senza che le Commissioni possano svolgere fino in fondo il loro ruolo. Si continua in un monocameralismo di fatto, che mortifica, a targhe alterne, un ramo o l'altro del Parlamento. E non si capisce per quale motivo non si dà la facoltà ai parlamentari nell'esercizio delle proprie funzioni di svolgere questo ruolo fino in fondo. Noi capiamo bene che siamo al cospetto di un Governo che è un gigante dai piedi d'argilla. Lo certifica il fatto che sul milleproroghe, in Commissione alla Camera, il Governo è stato battuto quattro volte. Lo certifica il fatto che la scorsa settimana, qui in Aula, il Governo è stato battuto tre volte con un livello di confusione continua. Noi di Fratelli d'Italia, con il nostro *leader* Giorgia Meloni, avevamo detto che non è possibile dar vita a esperienze di Governo in cui si mettono insieme le mele con le pere. Quando si arriva a dover scegliere e decidere secondo degli orientamenti ideali e delle convinzioni concrete, questo è il risultato: un conflitto continuo, che la nostra Nazione paga attraverso la mortificazione del ruolo del Parlamento. Non è possibile, poi, vedere il Presidente del Consiglio che si irrita e richiama tutti dalla libera uscita. Se il metodo Draghi dell'ultimo anno di Governo dovesse essere quello della minaccia permanente delle dimissioni nel cassetto, allora - carissimi colleghi - il consiglio è che, se c'è tanta fretta di andare a casa il giovedì, sarebbe stato molto meglio tornare al voto. Gli italiani vi avrebbero accontentato in maniera molto lieta. Ad ogni buon conto, giusto per rivendicare qualche risultato che la dice lunga sul nostro modo di intendere la funzione di opposizione, anche in questo provvedimento Fratelli d'Italia ha portato molte proposte. Alcune delle proposte della maggioranza, peraltro, sono proposte che ci avete bocciato su altri provvedimenti, a dimostrazione che siete anche capaci di sottrarre con poca destrezza quello che è il lavoro compiuto dagli altri. Ci piace sottolineare il risultato che abbiamo ottenuto con l'approvazione di un emendamento che ha innalzato il tetto dell'utilizzo del contante da 1.000 a 2.000 euro. Si tratta che darà un po' di ossigeno e la possibilità di rilanciare un po' i consumi; quei consumi che avete distrutto attraverso la scelta scellerata dell'utilizzo del *green pass*, una misura che è servita assolutamente a nulla, soltanto a limitare le libertà individuali. Non ha avuto alcun effetto concreto dal punto di vista sanitario, ma è stata devastante dal punto di vista economico.

- ognuno vive nel proprio mondo, ma ci sembra che il mondo non viva in ognuno di noi. Quindi, se avete l'occasione, in questo ultimo anno, dimostrate, con un guizzo di dignità e di orgoglio, che il Parlamento non è il passacarte del Governo.

è difficile oggi intervenire in Aula su un provvedimento così importante, dopo quello che è accaduto questa notte, con le parole importanti e unitarie che sono state dette questa mattina in Senato sulla guerra in Ucraina. Ci troviamo davvero a discutere e ad approvare in quest'Aula un provvedimento che ormai è diventato parte integrante della stessa nostra attività parlamentare. Mi preme soffermarmi qualche momento su una questione preliminare, che però attiene al nostro ordinamento nel suo complesso Già dal nome che viene tradizionalmente attribuito al provvedimento che siamo chiamati a esaminare oggi ("decreto milleproroghe") emerge la vastità e l'ampiezza degli argomenti che vengono toccati. Il decreto milleproroghe è uno strumento che nasce dalla necessità di porre parziale rimedio a quell'instabilità e a quell'incertezza che sono intrinseche nel nostro ordinamento. Mi pare evidente che un simile strumento, che dovrebbe servire come *extrema ratio* e in via eccezionale, sia da anni utilizzato in maniera sistematica, lasciando peraltro inalterati quei problemi che attanagliano da troppo tempo il nostro sistema sotto il profilo istituzionale e soprattutto legislativo. L'essenza di questo provvedimento ci dimostra che è necessario che Parlamento e Governo si facciano portavoce di una maggiore compiutezza e certezza verso quel complesso di norme che, per quanto essenziali e attese, non possono rimanere nell'incertezza ed essere prorogate di anno in anno. Sono consapevole che questo lavoro difficilmente potrà essere compiuto nella coda finale della legislatura, ma ci tengo, anche a nome del Gruppo che rappresento, a sottolineare la necessità di un cambiamento in meglio sotto questo specifico profilo, affinché non si debba sempre ricorrere allo strumento del milleproroghe senza avere una visione d'insieme complessiva. Al di là di queste riflessioni preliminari, credo comunque che il decreto-legge in esame contenga risposte molto positive e importanti nei confronti di un ampio ventaglio di criticità e di questioni che il Governo ha affrontato in prima battuta e che il Parlamento, in fase successiva, ha integrato e migliorato, nell'ottica e nel solco dei compiti che la Costituzione ci affida. Su questo specifico aspetto tornerò in maniera più puntuale alla fine del mio intervento. Desidero intanto sottolineare l'impegno che le Commissioni I e V riunite alla Camera hanno manifestato nel concludere un provvedimento così ampio e trasversale. Ovviamente non posso non esprimere rammarico per l'impossibilità di analizzare e modificare in maniera puntuale il provvedimento anche in questo ramo del Parlamento. Credo in ogni caso che il lavoro dei colleghi e delle colleghe della Camera sia stato proficuo, anche grazie all'importante sponda che è stata offerta dai relatori del provvedimento, ma anche dallo stesso Governo, che ringrazio, e da tutta la maggioranza. Italia Viva-P.S.I. ha lavorato con grande intensità, lealtà e correttezza politica e istituzionale. Pur nella carenza sostanziale di risorse, credo che il lavoro svolto sia stato notevole e proficuo per gli importanti risultati raggiunti. Per ragioni di tempo, signor Presidente, non mi è permesso ripercorrere in maniera analitica le modifiche emendative che abbiamo proposto e che sono state approvate, ma proverò a concentrarmi su quelle più significative. Penso - ad esempio - alla proroga dell'applicazione delle disposizioni di semplificazione in materia di occupazione del suolo pubblico e delle aree pubbliche da parte dei pubblici esercizi, fino al 30 giugno del 2022, che ha consentito, insieme alla campagna vaccinale e al *green pass*, di mantenere aperti esercizi e attività. Penso anche ad un'altra norma, che riguarda i tanti giovani in cerca di occupazione per il settore dell'autotrasporto: si tratta della misura che consente ai giovani fino a trentacinque anni di età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali di fruire di un contributo per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'autotrasporto delle merci. Si tratta di risposte importanti e per questo voglio ringraziare i colleghi delle Commissioni di merito, che hanno operato anche in stretto contatto con il vice ministro Teresa Bellanova, che ringrazio. Voglio anche citare il lavoro, nell'ambito della materia dei trasporti, che ha portato all'approvazione di un testo che consentirà - da un lato - l'erogazione in favore del fornitore di lavoro portuale di un contributo fino a 90 euro per il lavoratore, anche per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, e - dall'altro - alle autorità portuali di destinare l'1 delle proprie entrate derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco proprio all'incentivazione del pensionamento anticipato dei lavoratori portuali. dunque tanti i contributi che Italia Viva-P.S.I. ha voluto dare come Gruppo parlamentare alla conversione di questo decreto-legge ed è questa la chiave di lettura con cui auspico si leggano tutti i correttivi che sono stati proposti durante il lavoro in Commissione. Il Parlamento ha il potere e il dovere di dare il proprio contributo nella fase di conversione di un decreto-legge adottato dal Governo. Voglio sottolineare questo aspetto soprattutto alla luce delle giornate particolarmente delicate in Commissione. Quando un Governo è sostenuto da una maggioranza così tanto ampia come mai si era visto, non vi è da stupirsi se le diverse sensibilità emergono nitidamente nel confronto parlamentare, magari su temi caldi e sentiti, ma questo rientra nella normale dinamica parlamentare. Al contrario, le diverse prospettive possono costituire un *plus* del dibattito, purché rimangano nei ranghi di un confronto e soprattutto purché non si metta in discussione il significativo percorso che è stato tracciato da questo Governo e che oggi noi non possiamo permetterci di disattendere.

Siamo stati i primi a chiedere un cambio di passo e per questo siamo stati anche duramente attaccati. Ora che, grazie al lavoro compiuto dal presidente Draghi e dalla squadra di Governo, finalmente stiamo andando nella giusta direzione, certamente non sarà Italia Viva-PSI a mettere in discussione la linea politica dell'Esecutivo, che noi sosteniamo fortemente e al quale vogliamo confermare e ribadire la nostra piena fiducia. A nome dei colleghi di Italia Viva-PSI annuncio, quindi, il nostro convinto voto favorevole.

un altro *vulnus* al bicameralismo e mi chiedo veramente cosa si voglia fare in futuro per evitare queste situazioni. Come ho spiegato già diverse volte, non è possibile che un ramo del Parlamento, che non solo ha il diritto ma anche il dovere di esaminare i provvedimenti governativi, non sia messo in grado di poterlo fare. Nonostante questo, il Gruppo per le autonomie voterà a favore del provvedimento in esame. Grazie anche al lavoro dell'altro ramo del Parlamento, il testo offre una serie di risposte ai cittadini, alle imprese, alle pubbliche amministrazioni impegnate nel percorso di uscita dall'emergenza. La più importante è sicuramente quella sul *golden power,* col mantenimento dei campi di applicazione estesi durante il Covid. Negli ultimi mesi abbiamo visto l'importanza di questa norma rispetto a interessi nazionali che vanno protetti e tutelati. Pertanto, non solo la proroga ma probabilmente servirebbe un intervento normativo che renda strutturale il ruolo dello Stato rispetto a settori e imprese che ricoprono un ruolo strategico. Vanno bene tutte le proroghe in materia fiscale; la riapertura dei termini per il pagamento delle cartelle rateizzate allo scoppio della pandemia; i sei mesi aggiuntivi per la restituzione dei prestiti garantiti dallo Stato fino a 30.000 euro; la proroga delle agevolazioni fiscali sull'acquisto della prima casa; la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori nel caso di domanda incompleta. Importanti sono anche le norme per le pubbliche amministrazioni; la possibilità per le Regioni e le Province autonome di anticipare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione anche per il 2022; la proroga per la stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione; l'anno in più per lo svolgimento dei concorsi pubblici in Ministeri, agenzie fiscali, forze di polizia e vigili del fuoco. Numerosi sono poi gli interventi a tutela dei settori produttivi, tra i quali quelli a favore dell'agricoltura, con nuovi termini per la revisione periodica delle macchine agricole e la proroga degli incentivi riguardanti gli impianti di produzione energetica alimentati a biogas naturalmente la proroga dei termini relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali e all'IVA per le imprese d'allevamento colpite dalla recente diffusione della peste suina. alle misure per l'autotrasporto, col bonus di 2.500 euro per i giovani tra i diciotto e i trentacinque anni che vogliano conseguire la patente per guidare il camion e favorire così un ricambio generazionale, anche per ragioni di sicurezza. Una menzione particolare merita il *bonus* per lo psicologo, perché ci ricorda che la crisi non ha avuto soltanto costi di natura economica o sanitaria; c'è una questione che attiene alle giovani generazioni che richiede grande attenzione e il *bonus* ha anche questo significato. Insomma, nella fase che stiamo attraversando, questo provvedimento ha assunto un ruolo ben più ampio di quello che generalmente occupa. Come dicevo, è diventato uno dei punti di risposta al percorso di fuoriuscita dalla crisi e, pertanto, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie

non è facile prendere la parola in un momento così drammaticamente difficile per il mondo intero. Noi stiamo parlando di un ridicolo decreto - e spiegherò

si sono spellati le mani per le parole usate in occasione dell'elezione del nostro Presidente della Repubblica non hanno lasciato passare che poche ore per andare di nuovo verso il voto di fiducia.

a una forma di Parlamento soggiogato, con un Governo che viene qui semplicemente per avere una formale autorizzazione a procedere, che non è quella prevista per i magistrati, ma quella che a noi in questo caso viene richiesto di dare. Nel merito, signor Presidente,

la proroga per l'abbassamento del tetto del contante, che quindi per quest'anno non passa a 1.000 euro, ma rimane a 2.000 euro; sarebbe stato davvero demenziale,

con tale misura facciamo anche in modo che quegli stranieri vadano a fare acquisti all'estero, magari nella confinante Austria, dove possono utilizzare il contante senza dover ricorrere ad altri mezzi di pagamento. Il risultato è quindi rivendicato con orgoglio da Fratelli d'Italia, mentre il Governo credo abbia ben poco da rivendicare. Il collega Steger, che mi ha preceduto, ha parlato del *bonus* psicologo. Nel merito sono d'accordo - ci mancherebbe

che il *bonus* psicologo è da addebitare all'incongruenza politica di chi ha voluto gestire la pandemia in questo modo vergognoso. Non sono il cittadino e la fiscalità generale a doversi assumere il costo del *bonus* psicologo, ma deve essere il Ministro che, imperterrito, con l'avallo del Governo, è rimasto al suo posto, continuando con una politica sanitaria che in tutta Europa non ha eguali

Ma non basta. Cosa avete fatto, signori del Governo, sul tema dell'energia? Come ho detto, siamo alle porte di una guerra che rischia di essere mondiale.

però, le aziende non riescono più a essere competitive sui mercati e le famiglie probabilmente non riusciranno più a scaldarsi. Vorrei capire dal MoVimento 5 Stelle se è il caso di chiudere anche il gasdotto TAP. Vogliamo bloccare anche il gas che viene dall'Africa? Almeno io ricordo che la posizione del principale partito di Governo era quella di chiudere la TAP per il passaggio del gas africano. modo, ricordo che il primo partito del Governo Draghi è contrario ai rigassificatori. Quindi, niente gas da stoccare. Dove è, allora, il Governo dei migliori? Qual è la risposta energetica che diamo al nostro Paese e all'Europa? Dove volete andare?

No, signori della maggioranza, voi non avete messo insieme il Governo dei migliori: voi avete messo insieme di tutto e di più per mantenere la poltrona, cosa diversa dal Governo dei migliori.

con la conseguenza che le nostre imprese idroelettriche non fanno da anni investimenti perché - logicamente - non possono contare sul tempo per poterli ammortizzare. *(Applausi)*. Questo significa

per cento di minor produzione energetica per colpa delle mancate proroghe, che noi non facciamo mentre la Germania, la Francia e gli altri Paesi europei fanno. È una vergogna e siamo stanchi, signor Presidente. Mi rivolgo all'unico rappresentante del Governo rimasto in Aula: dica al presidente Draghi che così non si può andare avanti.

Governo, colleghi e colleghe, siamo qui ancora una volta a fare una dichiarazione di voto sul decreto-legge di proroga termini, che potremmo definire ormai un decreto annuale, tutti gli anni siamo qui a snocciolare quali sono all'interno di questo provvedimento i tanti termini che vengono prorogati con un intento ben preciso, però, che è quello di far

l'invito che il presidente Draghi ha rivolto, anche nella sua conferenza stampa, per collaborare il più possibile. Il Parlamento è pronto a questo, lo sappiamo bene in quest'Aula e ce lo siamo detti più volte: che a tutti noi interessa è poter esaminare al meglio i provvedimenti, in modo da poter dare risposte il più possibile vicine e di vero aiuto ai tanti che possono essere in difficoltà.

ai provvedimenti che il Governo invia alle Camere. Ci sono altresì sicuramente la voglia, la volontà e il desiderio di esercitare appieno il nostro ruolo e il nostro dovere.

tutti i provvedimenti che in qualche modo sostengono e aiutano la vera ossatura di questo Paese, cioè i Comuni, soprattutto quelli piccoli, devono essere accolti. Credo che ci debba essere, anche nei provvedimenti a venire, grande impegno e interesse da parte sia del Governo, che deve avere grande attenzione - lo ripeto - soprattutto nei confronti dei piccoli Comuni che sono la vera struttura di questo Paese, anche del Parlamento. L'altro aspetto che sottolineo - vedo che ha interessato moltissimo anche il senatore De Bertoldi è sicuramente il *bonus* salute mentale. Permettetemi questa mattina di fare alcune precisazioni, perché credo che il sillogismo che sento usare da tanti e che ha usato anche il senatore De Bertoldi - che invito a rimettere la mascherina, peraltro - ovvero

sia causato soltanto da questi due anni di pandemia equivale ad affermare una cosa che non è vera. Sappiamo ormai da studi scientifici ben consolidati che il peggioramento di tante situazioni di disagio è progressivo negli anni, anche se certamente è innegabile che questi due anni abbiano dato un colpo finale a chi già viveva situazioni di difficoltà.

e che hanno bisogno non soltanto di un aiuto economico, ma anche di smontare quello stigma che ancora nel nostro Paese pervade e invade tutti coloro - non tutti ma tanti, veramente ancora troppi

tante volte viene consolato spronandolo ad andare a bere con gli amici e a parlare con loro. Ci sono dei momenti, invece, in cui soltanto i professionisti possono prendersi cura

molto importante è la scelta fatta dal Parlamento in relazione alla questione ILVA.

PMI e una serie di altre proroghe. Come hanno detto le colleghe e i colleghi che mi hanno preceduto, siamo in un momento molto difficile, gravissimo. Abbiamo tutti giustamente dichiarato che sosteniamo l'azione del Governo e del Presidente del Consiglio.

È il momento di rinsaldare le fila, di trovare aspetti di unità, non di scontro. La situazione che ci si presenta non è solo gravissima dal punto di vista della politica internazionale per il gravissimo atto di rottura

porrà problemi serissimi dal punto di vista della gestione e di quella che si era avviata come una crescita robusta del nostro Paese. Pensiamo solo alla situazione dell'autotrasporto, delle merci, che sta già procurando problemi serissimi. Penso ad alcune azioni che sono state poste in essere e mi rivolgo *in primis* ai colleghi della Lega; per esempio - agli emendamenti approvati contro il parere del Governo. Intendiamoci: il Parlamento ha piena autonomia ed è giusto che modifichi i provvedimenti del Governo, ma se siamo una maggioranza,

non ci possiamo giocare la partita con forzature e a colpi di maggioranza su questo o quel provvedimento, a prescindere da un'intesa comune sui passaggi che dobbiamo

Non è il momento della campagna elettorale. Spero che questo sia un elemento chiaro a tutti: così come vale per noi

Non ci possono essere azioni unilaterali di questo o quel partito. Spero che in un momento così difficile questo sia l'impegno di tutti i Gruppi.

Bisogna avere la capacità di costruire delle sintesi e essere tutti impegnati a portarle avanti. Infine, una piccola considerazione sul *bonus* salute mentale. è una situazione di emergenza e questo non può che essere un intervento straordinario nell'emergenza. Rimane però un punto strategico. I dipartimenti di igiene e salute mentale sono al disastro ed è indispensabile investire strategicamente su di essi. Da questo punto di vista, ribadisco quanto ho detto ieri: c'è bisogno di una riforma organica della sanità che sia in grado di interpretare il nuovo che ci impone il Covid-19 ed il nuovo che ci impone la situazione pandemica. che, nell'utilizzo di questo *bonus* si trovi un modo per costruire un rapporto tra l'utilizzo del *bonus* stesso e i dipartimenti di igiene e salute mentale,

non so se è chiaro - perché, essendo così delicata la partita, dobbiamo dire ai cittadini che utilizzano il *bonus* di capire bene da chi vanno e a quali capacità e a quali professionalità Noi dobbiamo stare molto attenti affinché una misura positiva non si trasformi in un *boomerang*. Concludo ribadendo un concetto politico. Troviamo il modo, come maggioranza, per cambiare anche il rapporto tra Governo e Parlamento, maggioranza e opposizione. però, dimostrare se siamo all'altezza del momento. E questo momento richiede unità, capacità di sintesi e capacità di lavorare insieme senza forzature e senza rotture.

è certamente complicato. È una giornata particolare. Ci siamo tutti svegliati di fronte a un momento storico che non avremmo mai voluto vivere: l'occupazione militare dell'Ucraina da parte delle truppe della Federazione Russa. Ovviamente, si pongono tanti quesiti e, quindi, parlare qui di un provvedimento denominato milleproroghe certamente non è il massimo.

attengono anche alla vita quotidiana di molte persone e alcuni dei colleghi hanno citato casi specifici. Tra l'altro, il provvedimento è stato profondamente modificato

ed evidente che talvolta converrebbe porre fine ai rinvii, ormai istituzionalizzati; molte questioni andrebbero definite,

decisioni che hanno un rilievo temporaneo, con un atteggiamento estremamente efficace e propositivo. Devo dire che i nostri colleghi deputati del Gruppo Forza Italia hanno inciso in modo determinante

patologicamente viziata, dalla pandemia. Di fatto il nostro sistema bicamerale - fatemi fare l'esponente della Commissione affari costituzionali fino in fondo

e questo ci ha impedito - visto che è stato votato alla Camera dei deputati soltanto l'altro ieri - di intervenire per migliorarlo ulteriormente. Noi di Forza Italia facciamo poca polemica. Siamo un partito che non riesce a essere di opposizione fine a se stessa. Siamo nati per migliorare questo Paese, siamo nati per governarlo, non siamo nati per cercare di utilizzare il malcontento e il mal di pancia delle persone e quindi per gratificarci del loro consenso, tra l'altro spesso velleitario e illusorio. Noi pensiamo a risolvere i problemi, pensiamo ad affrontarli, assumendocene la responsabilità, assumendoci la responsabilità delle scelte e talvolta anche a richieste che evidentemente contrastano con le esigenze nazionali del nostro Paese. Siamo una forza responsabile, siamo stati in tutti i provvedimenti che sono stati assunti da questo Governo, pur consapevoli di una maggioranza estremamente eterogenea che vede insieme partiti molto diversi tra loro. Ma, pur consapevoli di questo, siamo ovviamente altrettanto consapevoli del fatto che poi, alla fine, quello che sta a cuore a noi è fare del bene agli italiani, lavorare per il benessere del nostro Paese il benessere delle nostre imprese e delle nostre famiglie. *(Applausi)*. Questo significa anche avere uno spirito contraddistinto da concretezza, quindi poche chiacchiere, poco spazio ai mal di pancia: i mal di pancia cerchiamo di curarli, non di cavalcarli, non di stimolarli. Noi siamo contro l'antipolitica. Noi siamo contro il populismo, siamo contro le demagogiche posizioni assunte solo ed esclusivamente per prendere voti. Noi vogliamo prendere voti da quella parte d'Italia che è consapevole che i problemi devono essere affrontati e risolti anche e soprattutto governandoli, compartecipando alle decisioni. In questo milleproroghe ci sono alcuni di questi aspetti. Uno di questi - voglio citarlo prima di concludere - è stato a cuore, durante l'estate scorsa, anche a questo ramo del Parlamento, qui in Senato:

del provvedimento che fu assunto a suo tempo e che purtroppo, poi, non trovò un esito favorevole nel corso del mese di agosto 2021. In 2021. In questa occasione abbiamo invece colto l'obiettivo, con la promessa, da parte dell'attuale Ministro della giustizia, che finalmente si metterà mano ai provvedimenti legati alla geografia giudiziaria che troppo sbrigativamente erano stati affrontati e risolti tagliando e sforbiciando, senza intervenire in modo puntuale sui territori. Speriamo che in questo tempo sarà concesso di intervenire in Abruzzo, come in altre Regioni d'Italia, per migliorare la

di fiducia al Governo e continuerà ad assumersi fino in fondo le responsabilità per portare l'Italia fuori da questa crisi, nella speranza che il mondo intero possa vivere in pace i prossimi mesi e anni.

che ogni volta non finisce di stupirmi perché, in spregio di ciò che la Corte costituzionale ha più volte precisato - ma fa parte ormai del nostro diritto positivo di omogeneo ha ben poco. L'unico criterio tassonomico che accomuna le norme contenute nel decreto-legge milleproroghe è, appunto, la proroga di qualche termine. termini che afferiscono a materie completamente diverse. Ma - tant'è - ormai è un appuntamento consolidato. Sottolineare che forse non è il modo migliore di procedere nello svolgimento dell'attività legislativa - mi rendo conto - è esercizio ozioso. Il provvedimento in esame, tra l'altro, tanto per aggravare la valutazione negativa che in generale sul piano sistematico, non politico, ora e adesso, si può formulare, non è stato da noi quasi neanche letto; è arrivato come una meteora e come una meteora attraverserà quest'Assemblea. Noi lo voteremo sicuramente (facciamo parte della maggioranza). Noi tutti, però, dovremmo prestare prestare più attenzione a questo problema, a questo nodo istituzionale: un sistema bicamerale dove in alcuni casi le due Camere funzionano come perché una Camera serve a correggere gli errori dell'altra ed è un bene che ciò accada, ma in altri casi un ramo del Parlamento non serve a nulla perché si trova a dover ratificare alla cieca ciò che l'altra Camera si spera abbia fatto al meglio.

Particolare attenzione è stata riservata agli enti locali, che sono la parte delle istituzioni più vicina ai cittadini. È noto che la qualità della vita migliore si rinviene nei centri più piccoli e la Lega è attenta a questo profilo. Per esempio, partendo dalle Regioni, è stato approvato un emendamento, appoggiato da tutti i colleghi della Lega, volto al sostegno delle Regioni e delle Province autonome, mettendo a disposizione l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, ovviamente dopo l'approvazione del rendiconto e prima - sia chiaro - del giudizio di parifica. È una misura concreta, che si inserisce all'interno di un'azione politica già iniziata con la legge di bilancio. Come Gruppo Lega abbiamo anche presentato alla Camera un ordine del giorno in cui si chiedeva che lo stesso avvenisse per gli altri enti territoriali, quindi i Comuni, ossia la possibilità di mettere a disposizione l'avanzo libero, il e le risorse residue del 2020 e 2021 per renderle disponibili nel 2022. Questa richiesta è venuta con forza dagli enti locali. Inoltre, abbiamo prorogato al 31 marzo il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali. Questo emendamento dimostra una grande attenzione della Lega per l'attuazione del PNRR. Apro una parentesi per dire che è un brutto acronimo, così difficile da pronunciare, direi quasi cacofonico; potevamo trovare qualcosa di meglio, il nostro italiano lo avrebbe consentito. È una misura importante perché permette di dare anche ai Comuni la possibilità di predisporre un piano operativo per la messa a terra delle opere necessarie per i bandi del PNRR. Per la scuola, previsto sostegno al personale dei servizi scolastici: grazie ad un emendamento abbiamo dato la possibilità a tutti gli istituti di fare assunzioni a tempo determinato che permettano di avere una continuità di servizio

è stato raddoppiato il fondo a favore degli assistenti degli alunni con disabilità. Tale emendamento ha portato al raddoppio da 100 a 200 milioni di questo fondo fondo molto importante, che fornisce un servizio agli alunni che hanno le maggiori difficoltà e richiedono quindi un maggiore sostegno. Dico questo per sottolineare l'attenzione al principio costituzionale di solidarietà, uno dei principali argomenti politici della Lega. la pazienza di ascoltarmi ancora qualche minuto perché non credo sia il caso di andare avanti con un elenco di provvedimenti eterogenei, visto ciò che ho detto Mi preme approfittare di questa occasione per segnalare che, a margine dell'approvazione alla Camera della legge di conversione del presente la Lega ha ottenuto l'approvazione di un ordine del giorno, politicamente molto importante, che impegna il Governo ad accorpare le date dei futuri *referendum* alle date delle elezioni amministrative.

perché una prassi, solo perché è tale, non vuol dire che sia una buona prassi. Separare le date significa far calare l'attenzione dei cittadini sul tema referendario. Il *referendum* è uno strumento di democrazia diretta, voluto dai Padri costituenti ed è nostro dovere sollecitare, aiutare e accompagnare i cittadini a esercitare un loro diritto. Separare le date significa mandare un pessimo segnale, un segnale diseducativo. Noi siamo qui anche per indicare dei percorsi di crescita per il popolo italiano ed è un buon argomento quello di unire le date: significa dire agli italiani i *referendum* sono importanti, che vi devono partecipare perché è un loro diritto ma anche un loro dovere, perché l'esercizio dell'attività referendaria fa parte delle garanzie costituzionali a presidio della sovranità popolare. quindi che questo ordine del giorno sia tenuto nella più alta considerazione da parte del Governo. E faccio un rapido cenno solo al tema del risparmio, perché accorpare le date vuol dire far risparmiare allo Stato molti milioni di euro

Signor Presidente, colleghi, stiamo per approvare oggi un provvedimento che tradizionalmente serve a varare interventi diversi tra loro, ma urgenti e necessari. Era doveroso farne buon uso e cogliere l'occasione per lavorare al servizio dei cittadini e delle imprese, del diritto alla salute e del lavoro. Compatibilmente con lo spazio riservato al Parlamento per l'attività emendativa, ancora troppo compresso - e il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha lavorato con i colleghi della Camera per migliorare il testo dell'Esecutivo e raccogliere istanze dei territori come quelle riguardanti l'Ilva di Taranto: la tutela dell'ambiente e della salute sono diritti prioritari e irrinunciabili e da qualche settimana principio fondamentale della Costituzione italiana. Le bonifiche, pianificate e finanziate da tempo, sono diventate per noi improcrastinabili.

Non era possibile rinunciare alle tanto attese attività di risanamento ambientale per un imprecisato e indefinito processo di decarbonizzazione, di cui peraltro non si conoscono i contenuti dell'investimento, il fabbisogno finanziario, il piano industriale e molti altri elementi indispensabili. Inoltre, definanziare le modifiche avrebbe significato anche rinunciare definitivamente al possibile impiego degli oltre 1.200 lavoratori dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Non tutto è andato come auspicavamo e, soprattutto, secondo le necessità dell'Italia. Il *blitz* con cui è stata portata a 2.000 euro la soglia per i pagamenti in denaro contante va in netto contrasto con gli impegni e gli obiettivi fissati dal PNRR. In questo modo abbiamo innestato la retromarcia rispetto alla strada che avevamo intrapreso negli anni dei Governi Conte con il *cashback*, la digitalizzazione e la tracciabilità dei pagamenti. *(Applausi)*. Per noi non va bene. Secondo noi, il potenziamento degli strumenti di pagamento elettronici deve essere al centro del lavoro con cui stiamo costruendo l'Italia dei prossimi anni. Lo sviluppo digitale ha enormi potenzialità in termini di semplificazione e contrasto all'evasione che, come sappiamo, per l'Italia è un autentico macigno. Tuttavia, il lavoro positivo svolto su questo decreto-legge vanta altri risultati di cui render conto e che inorgogliscono il mio Gruppo. Abbiamo introdotto il *bonus* psicologo. Dopo lo stanziamento, previsto nell'ultima legge di bilancio, di 25 milioni di euro per i disturbi alimentari e il potenziamento del sostegno psicologico nelle scuole, siamo riusciti a portare a casa questa conquista. Si tratta di un aiuto concreto verso tutte le persone che si trovano a vivere un disagio che è ancora troppo un tabù e che invece sappiamo bene quanto sia presente, ancor più dopo questi due anni di pandemia che hanno messo a dura prova i nostri equilibri. Il *bonus* arriverà a 600 euro nell'anno e potrebbe riguardare circa 18.000 persone. Abbiamo poi stabilito l'accantonamento, per l'anno 2022, di 32,5 milioni di euro destinati a strutture innovative e di qualità nell'erogazione di prestazioni pediatriche oncologiche. Mai come Mai come in questa fase è indispensabile destinare risorse alla cura e alla prevenzione. Tra le drammatiche conseguenze del Covid c'è anche la minore attenzione riservata alle altre patologie. Dopo una battaglia andata avanti per mesi e l'interlocuzione con il Governo e nella maggioranza, è stata finalmente approvata la proroga per mantenere aperti i tribunali abruzzesi. La proroga prevede di differire di un anno la chiusura delle sedi dei tribunali abruzzesi di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano al fine di revisionare e aggiornare il modello della geografia giudiziaria. In Commissione giustizia al Senato un apposito disegno di legge del MoVimento 5 Stelle prevede un riordino complessivo della dislocazione dei tribunali in Italia per porre rimedio a diverse storture prodotte dalla riforma del Governo Monti varata nel 2012. A dieci anni di distanza è opportuno evidenziare come quel provvedimento non abbia raggiunto gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione che si poneva e come abbia al contrario prodotto notevoli criticità, lasciando grandi territori nel nostro Paese privi dei necessari presidi di giustizia e legalità. Infine, voglio ricordare che, grazie a un emendamento approvato in Commissione bilancio alla Camera, gli enti di ricerca pubblici potranno proseguire con le stabilizzazioni del personale anche nel 2022. Il Consiglio nazionale delle ricerche, in particolare, potrà utilizzare 10 milioni di euro stanziati nella legge di bilancio 2022 per assumere i ricercatori anche quest'anno. Presidente, per tutte le motivazioni elencate, il MoVimento 5 Stelle voterà a favore del provvedimento in Signor Presidente, lei ha ragione quando dice che l'ululato non è una forma di dissenso consono a quest'Assemblea, così come certamente non lo è il lanciare carte sulla testa del Ministro che annuncia l'apposizione della quarantesima questione di fiducia alla Camera.

che ripetiamo le stesse parole in un depauperamento delle parole stesse. Eppure, non è cosa meno grave. C'era un tempo in cui, anche in TV, si declamava la bellezza della nostra Carta costituzionale come la più bella d'Europa. È difficile modificare la Costituzione: c'è un articolo specifico che stabilisce come, in che modalità e con quali

Questa vi appare cosa da poco ma non lo è, perché stiamo perdendo la nostra struttura democratica dettata dalla nostra Costituzione, che è la prima legge su tutte le leggi. *(Applausi)*. struttura architettonica che ci rende una Repubblica bicamerale e così avviene che, a fine febbraio, ci troviamo con un'ennesima questione di fiducia a ratificare ancora un

come ha detto la collega, dati agli enti preposti a mettere in atto le leggi, possono essere e sono già comprese nelle leggi stesse...

Grazie,

Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'Emiciclo. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(È

Signor Presidente, oggi ricorre un anniversario di grande dolore per il popolo azerbaigiano: si ricordano infatti i trent'anni dal grandissimo eccidio di Khojaly, commesso dalle forze armate dell'Armenia contro i civili azerbaigiani nella città di Khojaly in Azerbaigian. Ciò che è accaduto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 1992 rappresenta una delle pagine più atroci della storia contemporanea, un grande crimine commesso contro la popolazione civile azerbaigiana durante i decenni del conflitto con l'Azerbaigian, la pagina più tragica nella prima guerra del Karabakh: 613 persone, tra cui 63 bambini, 106 donne e 70 anziani, vennero brutalmente uccise; 1.275 persone furono fatte prigioniere, tenute in ostaggio e torturate. Il destino di altre 150 persone rimane ancora sconosciuto; famiglie sterminate e bambini orfani di entrambi i genitori. La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella decisione del 22 aprile 2010 inerente ai crimini commessi a Khojaly, giunse a un'importante conclusione, valutando il comportamento degli autori delle atrocità commesse come atti di particolare gravità equiparabili a crimini di guerra o crimini contro l'umanità. Vorrei sottolineare che ancora oggi gli autori del terribile massacro restano impuniti ed è di grande importanza, ancor più in un momento così drammatico come quello che viviamo a livello mondiale, che la comunità internazionale insista perché vengano riconosciute le responsabilità di questa strage e l'Armenia chieda perdono per quanto compiuto, interrompendo definitivamente la catena dell'odio, permettendo una reale conciliazione tra i Paesi e la normalizzazione della regione.

la fiducia che abbiamo appena approvato, posta sul decreto cosiddetto milleproroghe, mi rende quasi necessario sollecitare la risposta ad alcune interrogazioni che avevo già presentato in precedenza e che hanno come oggetto la tutela della salute attraverso attraverso quello che io considero uno dei determinanti di salute più importanti che ci sono. Quando si entra nel Ministero della salute, i determinanti di salute evidenziati sono quattro

per cui fino a poco tempo fa consideravamo la Philip Morris, nella sua comune scoperta o perlomeno nella sua proposta commerciale del tabacco riscaldato, come in fondo l'equivalente di una grande azienda produttrice che, non potendo investire adeguatamente - anche perché in Italia è ancora vigente la legge Sirchia su questo punto - inventa un prodotto inventa un prodotto che è il tabacco riscaldato. Lo fa impiantando un'azienda molto grande in Emilia Romagna e, quindi, mettendo in gioco una serie di posti di lavoro che dovrebbero fare da copertura al danno esplicito alla salute che il tabacco comunque cagiona. Pochi giorni fa

la quantità di nicotina nei confronti della quale ha contratto assuefazione. Anche questa è un'aggressione alla salute; anche questo viene dalle grandi aziende; anche di questo ci rendiamo in qualche modo complici. Vorrei avere risposta a dette interrogazioni, perché nel momento in cui la salute diventa un bene prezioso, nel momento in cui come ieri votiamo una norma che mette in relazione l'azienda e il bene salute e lo facciamo all'unanimità, l'idea che due delle grandi produttrici di tabacco trovino la massima collaborazione ai limiti della connivenza su prodotti che del tabacco sono la diretta emanazione a me sembra profondamente contraddittorio. Sollecito pertanto la risposta alle mie interrogazioni,

per sostenere questo settore che è stato colpito da una crisi energetica che si riverbera su tutti i cittadini, come vediamo dai rincari delle bollette. Per la terza volta in pochi mesi il nostro Governo ha stanziato miliardi di fondi pubblici per alleviare le sofferenze economiche di tutti i cittadini stessa cosa sta succedendo negli altri Paesi europei. L'Europa oggi si trova a essere epicentro di una crisi energetica su scala globale. Spiace, però, avere cognizione che in questa crisi energetica, per cui tutti i cittadini

soli a far fronte a questa crisi energetica. Ricordiamoci che siamo qui per fare gli interessi dei cittadini e non delle singole aziende di determinati settori energetici. *(Applausi)*.

nuova finestra"). Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che domani, alle ore 12,30, si terrà, con trasmissione diretta televisiva, un'informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sul conflitto tra Russia e Ucraina. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti, a eccezione dei Gruppi Misto e Fratelli d'Italia, ai quali sono stati attribuiti dieci minuti. Martedì 1° marzo, alle ore 10, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. L'intervento e la replica del Presidente del Consiglio dei ministri e le dichiarazioni di voto avranno luogo con trasmissione diretta televisiva. I Gruppi potranno intervenire in discussione generale per dieci minuti ciascuno. Seguiranno le dichiarazioni di voto sugli eventuali strumenti di indirizzo presentati. **Atti